definitivamente stabilito né che il sistema di elezione del Senato debba essere diretto né che debba essere indiretto, convinto, come sono, che sarà la discussione parlamentare

sostituendo le parole da «ed elette» fino alla fine con le seguenti: «e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini», proprio per tener aperta anche questa possibilità.

confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento definito dalla Costituzione», che mi sembra possa raccogliere anche il consenso dei presentatori.

in questo caso, il parere sarebbe favorevole

nostro a buon titolo, in quanto reca non solo la mia insignificante firma, ma quella di 40 parlamentari del Popolo della Libertà in sede di confronto, al quale ci eravamo detti del tutto disponibili, è stato sostanzialmente svuotato come un'arancia a cui si lascino soltanto gli "acinuzzi", signor Presidente.

Inoltre, non bastando, abbiamo accettato altresì di rimaneggiare largamente il punto *f)*, con una dizione che mi permetto di rileggere integralmente - perché a questo punto anche la parola si va piluccando dovrebbe essere, giusta le intese e non secondo i *desiderata*: «conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di piena sovranità legislativa democratica e e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini». Abbiamo dunque mollato pressoché su tutta la linea, nonostante che molti colleghi della maggioranza e delle opposizioni e delle opposizioni - ci abbiano incoraggiati, pregati, sospinti a mantenere la sostanza dell'ordine del giorno medesimo. Ciò nondimeno, siccome noi altri - e men che meno io, perché nessuno mi ha nominato sindacalista del Senato - non possiamo mettere in crisi un *iter* approvativo di un'importante riforma quale quella che si deve licenziare stasera, nè tampoco minare la stabilità di Parlamenti e Governi, e Governi, ci siamo adattati ad accettare questa formulazione della buccia e degli acinuzzi. A fronte di ciò, i nostri contraddittori non intendono,

A fronte di tutto ciò, cosa vi debbo dire? Eravamo al punto di non menare scandalo se di fronte a questa entrata a gamba tesa sulle riforme istituzionali la Presidenza, valutando l'esito del dibattito,

Neanche questo va bene! E allora, signori - io non posso provocare, perché non sono l'ultimo arrivato, né i miei 40 colleghi intendono destabilizzare nulla - se credete, vogliate approvare la buccia e gli acinuzzi del nostro povero ordine del giorno per riaffermare almeno la dignità del Senato in questo processo di interlocuzione di riforme che si va a mettere in moto. Dopo, poi, fate quel che volete dell'ordine del giorno G104, che credo seguirò dall'esterno dell'Aula, ma vi dico: resti la piena sovranità morale del Senato e di ciascuno dei suoi membri, perché si tratta di meri auspici. Quando affronteremo la materia, ognuno sarà libero di sostenere quel che vuole; per quanto mi riguarda, con il limite che il Parlamento è fatto di Camere sovrane, elette dal popolo e nella pienezza dei loro poteri legislativi, e su questo spero di non restare solo.

delle realtà popolari; *b)* conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di piena sovranità legislativa democratica e quindi elette

Presidente, accetto la formulazione proposta dal Governo. Faccio rilevare al senatore Benedetti Valentini che tutti, nell'esame di questo provvedimento, abbiamo abbiamo accettato anche delle soluzioni che non coincidevano totalmente con il nostro pensiero e con la nostra posizione politica. Tuttavia, io accetto

penso che, nella sostanza, l'ordine del giorno mantenga i contenuti per i quali era stato presentato.

nella legge sul federalismo fiscale, ma che neanche il relatore ha avuto modo di illustrare quei piccoli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati

ha permesso ai colleghi della Camera, in sede di princìpi generali, quindi nell'articolo 1, di affermare le norme generali del disegno di legge sul federalismo fiscale hanno diversi obiettivi, alcuni dei quali sono ovvii ed altri sono specificati meglio. Si è inoltre

dell'articolo 119 della Costituzione, improvvisamente, nei princìpi generali, si dichiara che vi sono anche norme generali sull'ordinamento della capitale, anche di tipo finanziario. Non c'è quindi la previsione sull'ordinamento finanziario, come sarebbe logico e coerente, ma c'è un discorso sull'ordinamento e - si aggiunge - anche di tipo finanziario.

colgo l'occasione, incidentalmente, per riferire un episodio che credo l'Aula abbia il diritto di conoscere,

il capogruppo della maggioranza capitolina Dario Rossin, collega del senatore Cutrufo qui presente in Aula, ha dichiarato che con il disegno di legge che stiamo per approvare a Roma viene riconosciuto il rango di Stato nello Stato.

e indirettamente anche il sindaco di Roma provvedano a smentirle categoricamente.

con l'emendamento 2.11 proponiamo di aggiungere alla fine del comma 6

della necessità di considerare le disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali. In pratica, non facciamo altro che riprendere il ragionamento svolto stamattina dal collega Bianco relativamente al fatto che nel provvedimento in esame manca la Carta delle autonomie locali.

Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nello scorso mese di dicembre,

Per questa ragione l'emendamento fu trasformato in ordine del giorno, approvato da quest'Aula in sede di prima lettura.

per il motivo per il quale abbiamo discusso, anche adesso, i vari ordini del giorno, cioè la necessità di non tornare ad una quarta lettura alla Camera. L'atteggiamento dell'opposizione è quindi fortemente contraddittorio su questo specifico punto, che fissa in modo chiaro e netto gli effetti che dovranno determinarsi attraverso l'applicazione del federalismo fiscale sull'andamento della pressione fiscale in Italia nei prossimi anni e sulla conseguente necessità l'obiettivo finale del federalismo fiscale sia quello di dare ai cittadini più servizi, migliori servizi e più controllo, secondo le responsabilità

il precedente ordine del giorno impegnava il Governo ad indicare il profilo di riduzione della spesa pubblica corrente e della pressione fiscale nei Documenti di programmazione l'attuale ordine del giorno impegna il Governo a fare questo con chiarezza e trasparenza nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria che dovrà essere presentato entro la fine di giugno. A questo punto vorrei che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, chiarisse la sua posizione e spiegasse a quest'Aula perché ciò che a dicembre è stato oggetto di minaccia di ostruzionismo sull'intero provvedimento

che si dica con chiarezza ai cittadini italiani che il federalismo fiscale è lo strumento che consente di avere uno Stato e i vari livelli di governo di migliore qualità e ad un costo finale per il contribuente che negli anni deve ridursi secondo un percorso certo e credibile.

che in sede di attuazione di questa legge si tenga fede al dettato legislativo e che il federalismo fiscale si realizzi davvero senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi, impegniamo l'Esecutivo a precisare «i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse».

in tutta la discussione sul federalismo, sull'esigenza di dare più trasparenza e più concretezza ai fattori di costo, di finanziamento e alle modulazioni con cui si passerà, opportunamente, dalla spesa storica alla spesa parametrata per standard e fabbisogni, in modo da garantire il finanziamento del livello delle prestazioni essenziali e delle funzioni essenziali dei Comuni, ed anche di quelle definite non fondamentali. Riconosco che la discussione che c'è stata in prima lettura al Senato e poi l'ulteriore affinamento introdotto dalla Camera dei deputati hanno prodotto dei risultati oggi, nel testo che verrà posto in votazione, ci sono precisi vincoli che impegnano a corredare i primi e poi i successivi decreti attuativi con i doverosi profili delle implicazioni contabili, anche relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard definiti sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Questo è un risultato che riteniamo possa essere ascritto ad uno dei significativi contributi che abbiamo portato nella discussione, che hanno determinato il miglioramento del testo inizialmente presentato alle Camere. si doveva e si poteva fare di più. Questo non è un appunto rivolto al ministro Calderoli, neanche ai presidenti di Commissione, al relatore o alla maggioranza, che hanno lavorato con uno spirito e un atteggiamento di concretezza e di attenzione al dialogo con l'opposizione che noi riconosciamo: credo che i risultati siano lì a dimostrare che questo è un modo giusto di far funzionare le Aule parlamentari. se c'è qualcuno che andrebbe messo in castigo dietro alla lavagna è il Ministro dell'economia che, sì, qualche fugace passaggio l'ha fatto, ma

che si potranno fare solo dopo e a conclusione del processo; noi chiedevamo simulazioni su come si costruiscono i nuovi flussi finanziari a copertura dei trasferimenti che vengono soppressi in base alle opzioni indicate nel testo del provvedimento, per poterne valutare le implicazioni e le conseguenze, anche allo scopo di poter fare scelte più consapevoli e meditate circa anche il *mix*, la composizione di quel *cocktail* di entrate che dovranno essere poi dettagliate per conseguire il risultato di garantire la copertura della spesa e innescare il processo dell'autonomia finanziaria. Questa cosa si poteva fare,

Queste avrebbero probabilmente fatto emergere che il processo di composizione e di scomposizione delle entrate, da porre a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali

vi sarà un risultato virtuoso di quest'operazione, che consisterà in più efficienza, più responsabilità, più trasparenza, e questo è un fatto positivo nell'interesse della modernizzazione del sistema Paese e della spesa pubblica; ma il Paese di Bengodi ce lo dovremo sudare e ciò avverrà nella fase di attuazione, quella più delicata e critica, nella fase di transizione, del passaggio da un modello ad un altro. altro. Queste sono le ragioni alla base della richiesta di questo ordine del giorno, perché quanto non è avvenuto prima non si può più eludere

con i Servizi del bilancio di Camera e Senato che, secondo me, hanno più competenze per poter sviluppare questa elaborazione. Disporre di queste simulazioni è fondamentale nella fase preliminare alla definizione del primo dei decreti di attuazione: in primo luogo, perché vi sono margini di come sarà articolato il meccanismo di composizione del finanziamento del sistema che possono essere oggetto di confronto sulle soluzioni migliori da assumere; e soprattutto, perché emergerà il vero problema, che costituisce per me una preoccupazione e un cruccio (e dovrebbe esserlo anche per tanti altri che hanno fatto l'esperienza di amministratori locali), del governo della fase transitoria del passaggio dalla spesa storica alla spesa per standard e fabbisogni, con particolare riferimento alle realtà comunali e a quelle funzioni non fondamentali, che certo non saranno decisive per la vita delle persone, ma sono molto importanti per migliorarne la qualità

del giorno potrebbe determinare un'utile assunzione di responsabilità da parte del Governo e speriamo che in questo modo si possa continuare, al di là del fatto che noi manteniamo noi manteniamo un atteggiamento che punta meno sulla propaganda e più sulla serietà e sul rigore, un dialogo e un'interlocuzione che in questo periodo hanno prodotto risultati positivi nell'interesse generale del Paese.

riguarda il perfezionamento dei poteri della Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Con questo emendamento, di consentire alla Commissione di avvalersi della collaborazione di una già istituita commissione, operante presso il Ministro dell'economia, che ha la responsabilità di vigilare sull'attività dei concessionari della riscossione.

L'articolo riguarda le competenze legislative delle Regioni, le conseguenti competenze amministrative e le relative modalità di finanziamento. l'emendamento 8.5 noi proponiamo di ripristinare il testo originario che avevamo approvato al Senato. Proponiamo inoltre un'integrazione, che peraltro è stata ampiamente discussa in questa sede: collocare l'intero trasporto pubblico come competenza regionale finanziata sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel testo emendativo che qui proponiamo torniamo ad inserire le funzioni e le competenze inerenti il diritto allo studio e, per quanto riguarda la materia dell'istruzione, torniamo ad inserire un riferimento all'intesa Stato-Regioni sull'istruzione, che può determinare un ampliamento delle competenze regionali in materia di istruzione proprio sulla base di questa intesa di carattere generale.

includere in questa competenza anche tutte le funzioni relative al diritto allo studio. Mi riferisco alla possibilità di accesso all'istruzione per tutti i ragazzi e alla possibilità di un adeguato successo scolastico e formativo per tutto il percorso dell'obbligo.

il federalismo mi sono speso, ho lottato nella mia vita per uno Stato delle autonomie, non sono mai stato un amministratore che ha pesato sulla disamministrazione. Pertanto credo fermamente che questa sia una rivoluzione che dobbiamo assolutamente portare avanti. Signor Ministro, stia attento agli ipocriti che le stanno vicino. Noi porteremo sempre porteremo sempre avanti la battaglia per far sì che il federalismo, come mezzo, sia strumento di un'amministrazione chiara ed efficiente e porti soprattutto

uno Stato moderno si costruisce non sulle furbizie, ma su regole che chiediamo ai pubblici amministratori e ai cittadini di rispettare.

mi vien da dire che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Ho cercato più volte di spiegare il fondo perequativo interviene per colmare il *gap* che esiste tra le risorse dell'autonomia impositiva dell'ente locale, della Regione, rispetto al fabbisogno standard.

a partire dall'entrata in vigore dell'attuale Testo unico sulle autonomie locali si è realizzata nel nostro Paese una interessante sperimentazione. Molti Comuni di piccole dimensioni si sono consorziati in unione di Comuni e hanno gestito in modo unitario alcuni servizi pubblici per i quali è riconosciuto un principio di adeguatezza per cui è preferibile che vengano gestiti da una comunità più numerosa di quella composta da alcuni singoli Comuni. Sono alcune centinaia le unioni di Comuni che hanno

un approccio di tipo draconiano, ma che sia prevista la possibilità di incentivare adeguatamente i Comuni a gestire tali funzioni in modo associato.

correlata. Si tratta di affinare - questa è la proposta che noi avanziamo - le modalità con le quali si finanziano i servizi e le funzioni non fondamentali. Il disegno di legge sotto questo profilo non è garantista per i Comuni che possono non avere, per scarsa capacità fiscale, la forza per finanziare le funzioni e le attività non fondamentali. Questi tre emendamenti correggono tale impostazione che a noi non pare sufficiente del disegno di legge.

Senatore Franco

riguarda una norma che valutiamo con un giudizio molto critico rispetto a questo disegno di legge. Senato, già in prima lettura - e la questione è stata poi ulteriormente aggravata dalla Camera dei deputati - ha deciso inopinatamente di inserire nel disegno di legge delega sul sul federalismo fiscale la questione relativa alla disciplina, sia pur transitoria, delle Città metropolitane, ed ha fatto analoga scelta per quanto riguarda Roma capitale. Si è trattato di un di un compromesso politico, perché alcune forze politiche hanno voluto assolutamente che fosse così fatto. Naturalmente, la sede propria per normare in materia di Città metropolitane era quella del Codice delle autonomie.

certamente bellissima e di grande rilievo e importanza nella storia del nostro Paese, ma che non è mai stata considerata da alcun atto normativo come una Città metropolitana. Con un colpo di mano politico, Reggio Calabria è stata inserita nell'elenco delle Città metropolitane, sulla base di una valutazione di carattere, lo ripeto, esclusivamente politico. Noi consideriamo con la dovuta attenzione la città di Reggio Calabria, per ragioni che sono evidenti. Quando si è trattato, ad esempio, in una situazione molto delicata, di spostare nella prefettura di Reggio Calabria il coordinamento, ai fini del contrasto della criminalità organizzata, delle prefetture della Calabria, il Partito Democratico è stato in prima linea nel sostenere e nell'adottare quel provvedimento, che poi portò alla nomina del prefetto De Sena quale coordinatore dei prefetti della Calabria. quale coordinatore dei prefetti della Calabria. Siamo sempre disponibili a considerare la specificità e la delicatezza dei problemi di Reggio Calabria, ma, francamente, troviamo che risponda ad esclusive valutazioni di carattere politico l'inserimento di questa città in tale elenco.

Presidente, annuncio che voterò in dissenso dal mio Gruppo, anche perché penso che la città dello Stretto possa essere una risorsa per l'Italia.

*f)*, prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo

Roma ha delle specificità, che le vengono riconosciute, nel settore dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei beni culturali e quant'altro.

quasi pleonastico, va riconosciuto; per lo meno il Governo deve porre una certa attenzione su tale specificità della città di Roma per l'eccezionalità degli eventi e per la presenza di questa grande mole di turisti. In caso di interventi di carattere sanitario di emergenza, alla Regione Lazio non viene riconosciuto alcunché per la sua specificità. L'ordine del giorno G24.101, in maniera molto blanda, impegna semplicemente a valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse

Roma sostiene costi che non sono quelli previsti dalla quota capitaria per svolgere attività e servizi di emergenza nelle grandi manifestazioni del nostro Paese, del sindacato, della politica o connesse alla presenza del Vaticano.

Signora Presidente, colleghi del Senato, il Movimento per l'Autonomia ha avuto, sin dall'inizio del percorso politico, oltre che legislativo, di questo provvedimento, un atteggiamento di grande apertura rispetto a questa riforma del sistema della finanza pubblica, perché la considera il giusto preludio a un più importante provvedimento di riorganizzazione costituzionale dello Stato in senso federale. Questo perché noi abbiamo posto a fondamento della nostra azione politica il valore dell'autonomia, non solo territoriale ma anche culturale e politica, valore costituzionale. Inoltre, il nostro primo e più forte insediamento territoriale nasce in una Regione, la Sicilia, dotata di uno statuto costituzionale che sancisce il suo rango di Regione a Statuto speciale e, quindi, anticipatrice di un modello federalista, in quanto il rapporto tra Stato e Regione è un rapporto pattizio. Dobbiamo dolerci delle tante occasioni in cui questo rapporto è stato violato, sia per l'invasività del potere centralista dello Stato, sia per l'insipienza e l'ignavia dei rappresentanti politici regionali, che non hanno mai posto a fondamento della loro azione il valore dell'autonomia e sono stati soccombenti rispetto a questa invasività del potere statuale. Il tema che è stato poi evocato in contrasto a questo processo di riforma federalista spesso è stato quello della minaccia all'unità nazionale, come se questo processo disgregasse una unità nazionale della quale noi non rinveniamo traccia se non in una falsa retorica. Questo è il Paese europeo che annovera al suo interno le regioni più ricche del continente e le più povere, con un divario drammatico sia nella dotazione infrastrutturale, caro signor Ministro per le infrastrutture, che nella qualità dei servizi, nel reddito pro capite e nell'incidenza delle imprese che agiscono sul territorio. una differenza drammatica, alla quale 150 anni di falsa retorica dell'unità nazionale non hanno posto alcun rimedio, certamente anche per colpa di una cultura centralista che ha impregnato lo Stato, le istituzioni e le forze politiche. Nessuno ha posto rimedio in modo convincente a questa condizione. Questo Governo ha assunto su di sé l'impegno, nel quinto punto del programma di coalizione, di avviare una serie di interventi strutturali per il recupero di tale divario.

da quelle destinate al Mezzogiorno, sia attraverso i fondi FAS che attraverso i fondi strutturali, per finanziare gli ammortizzatori sociali, costituisce una doppia ingiustizia per questo Paese: verso il Sud, che è stato privato delle risorse destinate per legge

Operiamo lealmente con il Governo ricordando questo impegno, richiamando la sua responsabilità e richiamando questa lealtà ai patti di coalizione. La nostra lealtà non è mai mancata in quest'Aula e mai mancherà, a prescindere da qualche invito giornalistico a riflettere sulla sostanza della lealtà politica. Aspettiamo dunque che il Governo rispetti i suoi impegni, a fronte della nostra responsabilità politica che discende da un patto elettorale che intendiamo confermare

quando si prefigurava un successo ampio del centrosinistra (e non una risicata vittoria), con l'approssimarsi di cinque anni di dura opposizione. Questa è la linea, questa è la coerenza del Movimento per l'Autonomia nei rapporti politici, ma anche nella fedeltà al suo patto con il territorio. Consideriamo il federalismo equo e solidale una risposta vera per costruire un'autentica unità nazionale; un federalismo che promuova una concorrenza virtuosa tra i territori e che si fondi sull'eguaglianza dei punti di partenza. Amici, occorre sgombrare il campo anche dalla banalità e dai luoghi comuni. È pur vero che vi è una differenza profonda nel prelievo fiscale tra le aree del Paese, ma ciò discende dalla profonda differenza del reddito che si produce in quelle aree. Sfido chiunque a contestare il dato che in nessuna area meridionale la quota di spesa pubblica trasferita dallo Stato a quel territorio sia superiore alla quota trasferita in una Regione del Nord:

Amici della Lega, sono convinto che la partita non si è chiusa oggi e che la sfida che il centralismo porterà all'iniziativa federalista cominci a delineare i suoi contorni più inquietanti. E il contorno più inquietante è il compagno di strada politico di questo processo di riforma costituzionale, vale a dire la riorganizzazione, sempre più forzata, del sistema politico attorno ad un bipartitismo che pretende di racchiudere in sé tutte le rappresentanze politiche, culturali e territoriali. Noi, come Movimento per l'Autonomia, abbiamo reagito a questa pretesa e confidiamo nella volontà degli elettori di dotarci della forza necessaria a difendere il valore dell'autonomia, della rappresentanza politica e culturale. Consideriamo l'autonomia la nuova frontiera, la nuova sfida politica nel Paese, perché autonomia si coniuga con partecipazione democratica. Se libertà vuol dire partecipazione - come cantava una straordinaria composizione di un artista unico, la cui compagna abbiamo l'onore di avere tra i colleghi di quest'Aula quest'Aula - la sfida del Movimento per l'Autonomia è una sfida di libertà, perché vuole assicurare la partecipazione democratica e la rappresentanza autentica dei territori. E questa legge elettorale per le europee, se da un canto soffoca la rappresentanza con un iniquo sbarramento, assurdo ed ingiustificato, dall'altro, attraverso il voto di preferenza, consente di ricostituire l'autenticità del rapporto tra eletto ed elettore, negata delle prassi insopportabili delle liste bloccate che in questi giorni si tenta di realizzare capziosamente, anche con alcuni meccanismi surrettizi. Anche questa volta noi assicuriamo al Governo il nostro voto favorevole al provvedimento, pur con le modifiche apportate alla Camera dei deputati. Ma la nostra fiducia, il nostro apprezzamento e il nostro sostegno sono scanditi da un di più di vigilanza attiva affinché il processo federalista avanzi, affinché il sistema centralista arretri, affinché si ricostituisca un nuovo rapporto tra rappresentanza e autonomie e affinché questo Paese, attraverso questo virtuoso percorso di innovazione, possa davvero innescare un processo di sviluppo che tenda a riassorbire il divario tra le diverse aree e a determinare, non già la retorica dell'unità nazionale, ma un nuovo patto civile e politico della comunità, che dia vita alla vera comunità nazionale.

Il nostro no è ancora più forte e convinto di prima, perché il vostro provvedimento è stato peggiorato alla Camera e torna qui in Senato carico di contraddizioni e di problemi irrisolti. Non basta, infatti, promettere che si ridurrà la pressione fiscale e si diminuirà la spesa pubblica: bisogna anche dimostrare che ciò corrisponde al vero. La verità è invece che questo provvedimento non serve né a contenere, né a razionalizzare la spesa pubblica. Come può essere credibile, infatti, un federalismo nel quale non si sa chi fa che cosa e nel quale non sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini italiani? un federalismo in cui le funzioni fondamentali degli enti locali sono definite forfettariamente? No, quindi, ad un federalismo «tanto al chilo», buono per tutte le stagioni, che costerà caro agli italiani, a quelli che stanno al Nord come a quelli che stanno al Sud; un federalismo senza numeri, del quale non si conosce nulla, e ciò che si conosce induce ad essere preoccupati; un federalismo così evanescente da essere affidato ad un numero elevatissimo di variabili: 12 tributi, 5 soggetti istituzionali che decidono, 11 criteri direttivi, 2 fondi statali, 8 procedure attuative. Ma come si fa a teorizzare l'anarchia fiscale e spacciarla per una grande riforma? Secondo voi i conti devono essere fatti dopo e non prima di affidare a Regioni ed enti locali così ampi poteri di spendere e di tassare: secondo noi è pura follia. Voi volete, per mero calcolo elettorale, una delega in bianco: ma quale credibilità avete per chiederla? Parlano per voi i numerosi provvedimenti federalisti che avete messo in campo in quest'anno di Governo: 140 milioni di euro per coprire i buchi del bilancio del Comune di Catania; 500 milioni di euro per coprire i buchi del bilancio del Comune di Roma; per non parlare del buco di 200 milioni di euro del bilancio del Comune di Palermo. Avete tagliato circa un miliardo di euro di entrate a tutti i Comuni italiani per darli a pochi e certamente non virtuosi Comuni. Avete fatto meglio e di più della «Banda del buco» e di Robin Hood messi insieme: non solo avete tolto ai Comuni buoni per dare ai Comuni spendaccioni, ma lo avete fatto rubando i soldi al Mezzogiorno, cioè saccheggiando a piene mani i fondi FAS. Per non parlare della mancata soppressione delle Province, chiesta da tutti a gran voce prima delle elezioni, e che oggi invece fate diventare importanti centri di tassazione e di spesa. Avete violato l'articolo 119 della Costituzione che vi obbliga a garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche delle Regioni e degli enti locali. Senza tale copertura, infatti, non vi è federalismo fiscale, perché non vi è certezza di entrata e di spesa. E che dire dell'impatto del vostro finto federalismo sul debito pubblico? Il vostro federalismo fiscale non ne parla e non dice chi deve farsene carico. Dal nostro punto di vista, è chiaro che lo Stato dovrà onorare il pagamento degli interessi sul debito e quindi non potrà ridurre la pressione fiscale. Pressione fiscale ed equilibrio dei conti pubblici fortemente compromessi dalla grave crisi economica, a tal punto che lo Stato sarà costretto a spogliarsi di quante più funzioni possibili, trasferendole a Regioni ed autonomie locali. Queste, a loro volta, saranno costrette a aumentare le tasse per coprire vecchie e nuove funzioni. Avete però parlato del patrimonio pubblico e della sua distribuzione territoriale. Ma il patrimonio dello Stato non è posto a garanzia del debito pubblico? Come si fa a trasferirlo più o meno massicciamente a Regioni ed enti locali senza sottrarlo a tale importante garanzia e senza trasferire quote proporzionali del debito al sistema delle autonomie? Il vostro federalismo fiscale, secondo recenti stime, potrebbe costare alle casse dello Stato fino a 100 miliardi di euro per la sola fase transitoria (che dura fino al 2016). È quindi legittima la nostra denuncia, secondo cui questo falso federalismo scassa i conti pubblici e rischia di aggravare la già difficile crisi economica del Paese. È come mettere altra benzina sul fuoco, perché un Paese in cui le famiglie non riescono ad arrivare alla terza settimana è un Paese che rischia di spaccarsi sulla ripartizione delle risorse, così come la volete fare voi. Avete la memoria corta, e questo è molto grave. Avete già dimenticato i guasti che la riforma costituzionale del 2001 ha prodotto nel rapporto tra Stato e Regioni. Avete dimenticato che quella riforma sbagliata ha avuto il solo effetto di far crescere tutti i livelli territoriali della pubblica amministrazione, alimentando le caste nazionali, regionali, provinciali e comunali di politici e burocrati. Noi abbiamo un'idea diversa del federalismo fiscale: competenze e funzioni chiare e nette dello Stato, delle Regioni e delle autonomie; un ruolo insostituibile dello Stato nella perequazione e nelle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale. Il superamento della spesa storica come elemento che regola i rapporti finanziari dello Stato con gli enti territoriali è condivisibile, ma il costo standard deve essere depurato solo delle inefficienze della pubblica amministrazione e non anche delle differenze territoriali, economiche ed infrastrutturali che ancora oggi dividono il Paese. Voi caricate la differenza economica tra costo standard e costo reale sui cittadini inermi, che non hanno alcuna responsabilità per le inefficienze pubbliche. Cittadini che mettete nelle mani di cinque livelli di governo diversi, pronti a tassarli indiscriminatamente. Con questo provvedimento scompare la unità giuridica ed economica del Paese, perché gli strumenti che garantiscono il riequilibrio economico e sociale tra Nord e Sud sono a copertura incerta, sfuggono alla decisione e al controllo dello Stato e del Parlamento e sono affidati agli interessi contingenti delle Regioni più forti. Con il vostro federalismo vengono meno tutti i sistemi di programmazione economica e si affida al potere discrezionale di quattro Ministri la decisione sulle infrastrutture di ogni genere e tipo. Delle Regioni a statuto speciale abbiamo ampiamente detto: con questo provvedimento se ne determina la cancellazione senza modificare la Costituzione. Un federalismo fiscale, quindi, che non serve a nessuno: non serve agli italiani, che oggi chiedono al Governo solo di uscire dalla grave crisi economica e occupazionale in cui si trovano; non serve al Sud, perché non gli garantisce pari condizioni per poter competere con il Nord; non serve al Nord, perché non gli darà minore pressione fiscale e maggiore stabilità finanziaria; non serve alla Lega, se non per questa campagna elettorale, visto che la genericità delle norme e la entrata in vigore ultradifferita (forse al 2016, ma è più probabile al 2020) le regaleranno una piccola e modesta vittoria di Pirro; non serve a sinistra, perché non è lisciando il pelo agli elettori leghisti che si riprenderà dalla sua profonda crisi di identità e di credibilità. Serve forse al Presidente del Consiglio, che ha già annunciato qual è il suo vero obiettivo, sostenendo il *referendum* elettorale: eliminare ogni forma di dissenso politico interno alla sua maggioranza e ogni forma alternativa di competizione politica. Cari amici della Lega, l'onorevole Berlusconi ha trasformato questo pseudofederalismo fiscale in una clava contro di voi. Da un lato, fa finta di accontentarvi con questo provvedimento; dall'altro, lavora ad una intesa a sinistra sul *referendum* per cancellarvi. E voi dovete stare zitti, perché il patto elettorale è stato formalmente rispettato e non avete di che lamentarvi. Cari amici del Partito Democratico, il vostro voto acquiescente sul federalismo fiscale (che noi rispettiamo anche se non lo condividiamo) non vi farà guadagnare punti. La vostra propensione all'accordo sul *referendum* elettorale rischia di indurvi in errore, consolidando quel finto bipartitismo che serve a rendere automatica e ripetitiva la vittoria del Popolo della Libertà. La delega in bianco chiesta da questo Governo serve solo a questo fine: ad un piccolo quanto significativo capolavoro politico in danno dei cittadini italiani. Noi dell'UDC abbiamo deciso di cantare fuori dal coro, facendo una vera opposizione a questo federalismo falso, pericoloso ed iniquo. Abbiamo detto no e continuiamo a dirlo a gran voce, perché non vogliamo avere un peso così grande sulla nostra coscienza.

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il progetto politico-istituzionale del federalismo fiscale ha come obbiettivo l'attuazione della Costituzione e ne dà una chiave di lettura più conforme all'evoluzione sociale, economica, culturale e legislativa. Ridefinendo entrate e spese si tracciano infatti i veri confini e i reali livelli di governo e di responsabilità, dal centro dello Stato al più piccolo dei Comuni. infatti una riforma che introduce cambiamenti radicali nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, prefiggendosi di diminuirne la distanza: parliamo infatti del godimento pieno dei diritti proclamati solennemente dalla Costituzione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, per quanto oggi rileva, senza distinzione di luoghi di residenza. Dunque, la ripartizione di risorse tra Stato, Regioni, Comuni e Province è una grande questione, forse la più spinosa e probabilmente una delle più rilevanti. Il metodo impostato dal ministro Calderoli, che ringrazio a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, si è concretizzato in una collaborazione leale e costruttiva in Parlamento, cioè nel luogo primario e per noi unico della rappresentanza politica e democratica del Paese. Il voto di astensione che il nostro Gruppo aveva espresso al Senato in occasione della prima lettura voleva rappresentare un chiaro e propositivo stimolo di proposta, volto al miglioramento del testo. Uno stimolo che ha portato all'incremento delle garanzie di uguaglianza tra i cittadini, di equità, di giustizia sociale, di rispetto dei vincoli di bilancio, di rafforzamento dei princìpi di responsabilizzazione di tutti i livelli di governo della Repubblica. Abbiamo il dovere di essere fiduciosi, perché è giusto esserlo in una legge che si attendeva da circa otto anni, indispensabile per applicare concretamente la responsabilità fiscale, in senso federalista, nel nostro Paese. un'aspettativa tutta da verificare sul piano della concretezza, attraverso il contenuto dei numerosi decreti delegati applicativi a cui viene fatto espresso rinvio. Certo, anche l'Italia dei Valori avrebbe voluto ulteriori ed importanti miglioramenti, ma le riforme - rispettato il principio sacrosanto di unità del Paese e di democrazia orizzontale e verticale dei diversi sistemi di governo - impongono impongono concessioni reciproche, perché il sistema chiede riforme condivise, non da adottare brutalmente a colpi di maggioranza e sempre senza stravolgimento della Costituzione. Tra i punti che più caratterizzano il testo, anche sotto il profilo delle novità sostanziali, sono da sottolineare: il principio della sussidiarietà fiscale, l'introduzione dei costi standard, la titolarità dei tributi, la perequazione, la previsione di un sistema di contabilità pubblica e unitaria e del suo sistema di controllo. Per il nostro Gruppo è stato poi importante l'ulteriore e ultimo accoglimento di due ordini del giorno: l'uno volto al monitoraggio costante e puntuale dei possibili costi che potrebbero derivare dall'attuazione della presente legge delega e l'altro volto ad integrare i contenuti sociali dei fondi perequativi in capo alle Regioni ordinarie. La scelta di un federalismo solidale e compatibile lo rende dunque diverso da come veniva tradizionalmente inteso fino a qualche tempo fa perché finalizzato a ricercare il giusto equilibrio tra efficienza e trasparenza delle prestazioni e la solidarietà che da sempre ha caratterizzato noi italiani. rappresentanti del Governo, colleghi, la efficace ed equa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione potrebbe essere metaforicamente associata ad una raffigurazione pittorica: il Parlamento, attraverso il provvedimento che stiamo approvando, ha fornito al Governo, che avrà il delicatissimo compito di redigere i decreti delegati, la cornice, la prospettiva, i pennelli, i colori, la tela su cui lavorare. Se il Governo avrà la cura di dipingere questo quadro con lo spirito realista di fine Ottocento, mirando cioè alla completa aderenza tra la rappresentazione artistica (i decreti legislativi) e la realtà (il disegno di legge che stiamo approvando), l'opera d'arte diverrà effettivamente straordinaria, innovativa e positiva per il Paese. I parametri concreti per determinare i costi standard sono ancora tutti da costruire, e quando ciò avverrà si dovrà tener conto di tutte le variabili, ministro Calderoli, della dimensione dei territori, degli enti destinatari, delle loro condizioni fisiche e socio-economiche e delle caratteristiche delle popolazioni che si renderanno destinatarie e beneficiarie dell'eventuale perequazione conservativa, garante dell'esigibilità dei diritti di cittadinanza per tutti e su tutto il territorio nazionale. Noi dell'Italia dei Valori scegliamo di sostenere questa innovazione e da oggi controlleremo con determinazione ferma per impedire al Governo di inserire nella cornice che il Parlamento oggi fornisce, dotata di paletti e di sanzioni, qualsiasi elemento di mortificazione degli elementi di legalità, trasparenza, responsabilità e solidarietà, valori che sono per noi imprescindibili in quanto possono rendere diversa e migliore la qualità delle amministrazioni e la qualità della vita dei nostri cittadini, di tutti i cittadini, di tutte e di ognuna delle singole parti del nostro Paese. La positività dei decreti sarà direttamente proporzionale al loro grado di fedeltà e coerenza con la legge delega approvata. Questo provvedimento e soprattutto il suo *iter* hanno dimostrato in modo evidente due elementi che voglio rimarcare in maniera puntuale: la responsabilità e la forza costruttiva dei Gruppi parlamentari dell'Italia dei Valori della Camera e del Senato, oltre che la conferma del valore assoluto che noi diamo alle decisioni parlamentari, e soprattutto la forza del dialogo costruttivo di cui sono capaci le opposizioni quando la maggioranza non cerca di prevaricare. Qui ed ora voglio ringraziare i colleghi del mio Gruppo per l'infaticabile e prezioso lavoro svolto su questo provvedimento di cui sono orgoglioso ed a loro È per questo che siamo impegnati ad approvare questa norma. Il senso del federalismo per noi dell'Italia dei Valori è il richiamo ai principi di responsabilità dei governi territoriali, lo dicevo in premessa. Abbiamo proposto, e la norma ora diventerà legge, che tale responsabilità fosse codificata tra i principi, oltre ad essere esplicitata, prevedendo sanzioni pesanti per gli amministratori spreconi, clientelari e bancarottieri, fino alla loro ineleggibilità alle cariche pubbliche. Non potrà e non dovrà essere più possibile che dopo sprechi e dissesti i responsabili restino impuniti e che i contribuenti di tutta Italia debbano pagare per quegli sprechi e per quei dissesti. Questa legge deve rappresentare una grande sfida per l'innovazione istituzionale del Paese, una sfida nel tempo, cioè nel vivo di una crisi economica globale, e nello spazio, vale a dire al Nord, come nel Mezzogiorno del Paese. Paese. Il federalismo fiscale, infatti, serve al Nord per meglio contribuire alla crescita omogenea del Paese ed al Sud perché venga demolito il luogo comune di un territorio, vittima dei suoi stessi sprechi e bisognoso di un assistenzialismo ormai intollerante. L'Italia dei Valori vuole mantenere viva e solida l'unità giuridica, economica e socioculturale della nostra Nazione e continuerà a lavorare perché tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza, possano godere di pari e di effettivi diritti e di pari dignità sociale, premesse ed essenza della nostra stessa democrazia. Per questo voteremo a favore di tale di tale legge; per questo, e non per favorire una parte politica, che pure tanto ha fatto per portarla all'attenzione, né per fare un favore al Governo, ma perché riteniamo che il nostro Paese meriti l'innovazione. L'Italia dei Valori accetta questa sfida e su questa sfida nei mesi e negli anni a venire vuole confrontarsi.

oggi stiamo per approvare un provvedimento che entrerà nella storia di questo Paese. Con il federalismo fiscale si innescherà un meccanismo che trasformerà la struttura di questo Stato. Gli effetti saranno visibili a tutti, cambieranno tante cose ed in meglio. Cambierà il sistema del prelievo fiscale, il modo di amministrare la cosa pubblica; soprattutto, la cosa più importante, si andrà finalmente una volta per tutte a smantellare l'impostazione centralista e assistenzialista di questo Paese. Un modo di amministrare che, ricordo a tutti, ha prodotto nel tempo il più alto debito pubblico d'Europa, uno dei più alti del mondo, una zavorra che ha frenato e frena ancora oggi l'intero nostro sistema produttivo. Daremo finalmente autonomia finanziaria ai Comuni, alle Province, alle Regioni: la giusta risposta ai tanti cittadini che non si fidano più di chi amministra i loro soldi da lontano, nei Palazzi, nel segreto, ma chiedono invece forme di governo più trasparente e più vicine a dove vivono. Tanto per essere chiari: i soldi che i cittadini pagano in tasse rimarranno sul territorio; non andranno più tutti a Roma e non ci sarà più qualcuno che da Roma deciderà come spenderli. Saremo finalmente padroni a casa Taglieremo così sprechi e burocrazia ed andremo a responsabilizzare anche gli amministratori pubblici: sindaci, presidenti di Provincia o di Regione che sprechino denaro pubblico saranno commissariati e non potranno più essere eletti. La finiremo così, onorevoli colleghi, una volta per tutte, con opere pubbliche iniziate e mai finite, con le assunzioni per voto di scambio, con ospedali e strutture sanitarie costruiti e mai utilizzati. Tutto questo secondo il sacrosanto principio mai applicato nel nostro Paese che chi sbaglia paga. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Stiamo parlando, onorevoli colleghi, di una vera e propria svolta, che va a coronare un percorso iniziato ancora nell'Ottocento da Carlo Cattaneo, per cui il federalismo non è solo il modo più efficace per amministrare lo Stato ma acquista il valore di una vera teorica della libertà, sulla base del principio che fuori dal diritto federale saremo sempre discordi ed infelici. Tesi riproposte negli ultimi decenni - è giusto ricordarlo da Bruno Salvadori e da Gianfranco Miglio e che sono state sempre portate avanti con forza e determinazione dalla Lega Nord e da Umberto Bossi. Sono questi gli ideali su cui si è fondato il primo programma politico nella storia della Lega, pubblicato su «Lombardia Autonomista» nel 1982, che proprio al primo punto riconosceva la necessità di superare lo Stato centralizzato con uno Stato federale, capace di garantire, tutelare e rispettare tutti i popoli che ne fanno parte. Questa battaglia noi della Lega Nord l'abbiamo iniziata da soli, con la stampa le televisioni e tutti i partiti della cosiddetta prima Repubblica contro, ce lo ricordiamo bene. Questa battaglia l'abbiamo fatta direttamente sul territorio, stando il meno possibile nei palazzi e il più possibile fra la gente. È così partita dal basso, dal popolo, una reazione sempre più forte, sempre più decisa, che ha di fatto cambiato radicalmente le cose. I partiti della prima Repubblica hanno perso, sono stati cancellati dal voto popolare, e quelli che sono nati hanno per forza di cose dovuto adeguare i loro programmi a questo nuovo sentimento popolare. Per questo voglio oggi ringraziare, a nome anche di tutti i senatori del mio Gruppo, i tanti militanti della Lega Nord *(Applausi che da anni, animati solo dalla loro passione, stanno combattendo per cambiare questo Paese. Scritte, volantini, manifesti, gazebo, incontri pubblici e feste sono serviti a far comprendere a tutti la bontà delle nostre proposte. Grazie a questo sforzo, queste idee sono uscite dai confini delle regioni del Nord per dilagare anche nel resto del Paese. Oggi anche al Sud vogliono cambiare. In tanti si sono stancati di un assistenzialismo fine a se stesso, sterile, improduttivo, che in molti anni non ha cambiato le cose. I tempi sono dunque maturi per una riforma che non andrà a dividere ma che farà ripartire l'intero Paese. Raggiungeremo così finalmente gli altri Paesi europei, che da tempo si sono strutturati in un sistema federale. Nel nuovo millennio, infatti, nessuno Stato è in grado di garantire, attraverso un'amministrazione centralista, l'efficienza dei servizi alla popolazione. Per questo motivo la Spagna, la Gran Bretagna, la Germania, il Belgio - ne cito solo alcuni - hanno avviato o consolidato un processo devolutivo come risposta all'esigenza di miglioramento delle *performance* del sistema pubblico. Un esempio è sicuramente la Catalogna, una regione europea dove a fronte di un elevato livello di decentramento fiscale si registra un'importante crescita economica, collegata ad un forte sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Perché, colleghi, federalismo vuol dire risparmio di risorse, meno tasse, servizi migliori ai cittadini, anche e soprattutto a quelli più bisognosi E diventa così ancora più importante approvarlo oggi, vista la crisi economica che stiamo vivendo. Per queste ragioni il federalismo fiscale lo possiamo considerare, senza ombra di dubbio, il provvedimento parlamentare più importante di questa legislatura. Un progetto che in molti non credevano possibile e che invece oggi diventa realtà. Lo voteremo, è giusto ricordarlo, dopo solo un anno di vita di questa legislatura. Il Senato si è insediato il 29 aprile del 2008, oggi è il 29 aprile del 2009: sono trascorsi solo 365 giorni, esattamente un anno, un record per una riforma così importante. Abbiamo dimostrato a tutti che questo Senato sa lavorare bene e in fretta. Questi dodici mesi sono stati però molto intensi: riunioni preparatorie, audizioni nelle Commissioni, dibattiti, discussioni, confronti, passaggi parlamentari; tutto si è svolto, cosa mai vista in Parlamento, in un clima di lavoro sereno e costruttivo, senza scontri e senza contrapposizioni muro contro muro tra le forze politiche.

i Presidenti delle Commissioni interessate, tutti i Capigruppo ed i parlamentari per il contenuto personale che hanno dato.

Ora bisogna continuare con l'approvazione dei decreti attuativi, con il codice delle autonomie e con le riforme costituzionali. Tutto ciò lo possiamo fare usando lo stesso metodo di lavoro che abbiamo adottato per questa riforma e che ha sicuramente funzionato: il metodo del dialogo e del confronto con tutte le forze politiche presenti, sia di maggioranza che di opposizione. Aboliremo così, tutti insieme, il bicameralismo perfetto, faremo nascere una Camera delle autonomie, un Senato federale, e andremo finalmente a ridurre il numero dei parlamentari: è quello che la gente ci chiede ed è ciò che faremo. Grazie alla Lega, questa sarà la legislatura del cambiamento e delle riforme.

dall'inizio della legislatura, di cui oggi festeggiamo l'anniversario, è riuscito ad approvare una riforma come quella del federalismo fiscale e a smentire, forse soprattutto in ragione della complessità, della stessa difficoltà tecnica e della portata di questa riforma, il verbo presidenziale (del Presidente del Consiglio, non del presidente Schifani) secondo cui l'unica possibilità di governare è per decreti‑legge e l'unica possibilità di riformare è a colpi di maggioranza. Il fatto è che - credo che questa considerazione sfugga in particolare ad una parte del Popolo della Libertà - sul federalismo fiscale è intervenuta una cooperazione politica, un convergere politico sempre esplicito e rigoroso, che ha fatto sì che il testo in esame sia di fatto molto distante dal testo e dall'impianto originario, abbia accolto molte delle nostre proposte e sia, in definitiva, un testo utile non solo per le Regioni ricche del Paese, ma anche per quelle che mostrano difficoltà. Sul merito non torno: il nostro relatore di minoranza lo ha già fatto ieri molto bene in Aula e più volte ne abbiamo discusso. È il punto politico del voto di oggi che io vorrei Come è potuto accadere che, partendo da quel testo, si arrivi oggi, in sei mesi, all'approvazione definitiva in un clima di non compiuta condivisione (noi ci asterremo, come è noto), ma certo di una intelligenza vera su questo testo? Forse per l'accanimento o, meglio, per la determinazione che ha mostrato la Lega, per questa sorta di *laissez faire* che il Presidente del Consiglio ha concesso all'alleato leghista, intravedendo o vedendo con chiarezza la valenza identitaria che al federalismo fiscale veniva attribuita dalla Lega? Certo, ma queste non sono le ragioni, bensì le occasioni. Le ragioni sono altre e direi che sono tutte, ma proprio tutte, indicative del fatto che in questo luogo politico, che è stata la discussione durata sei mesi sul federalismo fiscale, si mostrino alcune contraddizioni molto vistose che sono maturate e si sono mostrate oggi con molta evidenza all'interno della maggioranza. da una contraddizione, che è di pieno rilievo istituzionale e di grande valore politico, che riguarda il ruolo e le funzioni degli enti locali nel Governo del Paese; non solo, anche nel suo modello di sviluppo. Le questioni che abbiamo più volte affrontato in quest'Aula, quella relative all'ICI, quindi alla sottrazione ai Comuni di risorse importantissime per l'esercizio delle proprie funzioni e l'altra, che abbiamo condensato anche in un ordine del giorno a mia firma, che riguarda la variazione del Patto di stabilità, per consentire che i Comuni possano mobilitare risorse e quindi essere essi stessi fattori dello sviluppo, rappresentano una delle prime contraddizioni. A fronte delle politiche governative di abolizione dell'ICI e di penalizzazione dello slancio, delle possibilità degli enti locali, del loro ruolo nello sviluppo del Paese e nella codecisione rispetto alle alle scelte di governo, mi pare che questa prima contraddizione si mostri con ogni evidenza. Tuttavia, potremmo anche affrontare le incoerenze che si manifestano sul terreno delle riforme istituzionali. Oggi il Popolo della Libertà, ed in particolare il suo Gruppo parlamentare qui in Senato, ha mostrato il volto del conservatorismo delle classi dirigenti - per dirla con Gramsci - da cui deriva l'ostilità al Senato federale, contro tutto e tutti, anche contro molti voti già assunti delle Assemblee di Camera e Senato anche in legislature precedenti, e quindi l'ostilità per il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli enti locali nella determinazione delle politiche di governo. Dall'altra parte, coerentemente, le le proposte che di volta in volta vengono annunciate alla stampa e ai *media* dal Presidente del Consiglio mostrano un carattere fortemente neoautoritario e un impianto prettamente centralistico.

E la vicenda che si è svolta oggi sugli ordini del giorno è proprio emblematica di queste contraddizioni. Se volessimo dare un nome ai protagonisti della vicenda che si è svolta qui (faccio questa notazione perché so quanto il senatore Benedetti Valentini sia un appassionato cultore del teatro), potremmo dire che il ministro Calderoli è il personaggio che presta fede agli impegni presi: il buono, l'affidabile; il senatore Benedetti Valentini è il luminoso interprete del conservatorismo delle classi dirigenti; il presidente Gasparri (nella difficoltà che gli riconosco in maniera proprio sympathica) tenta la strada della sottovalutazione.

su una picca; è un pezzo dell'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione che noi volemmo e quindi in qualche modo è la condivisione di un'idea, di un assetto moderno dell'Italia, di una nuova destinazione dei centri di governo e di decisione, pertanto consacra quella riforma che noi volemmo e quell'impianto per il quale bocciammo al *referendum* la controriforma voluta dal centrodestra. Vorrei dire al collega Bricolo, che ha orgogliosamente rivendicato l'idea del federalismo contenuta sin dal primo programma della Lega, che anche noi abbiamo qualche antenato molto illustre: mi riferisco ad Altiero Spinelli; la nostra idea del federalismo parte da Ventotene. Il presidente Gasparri tenterà nel suo intervento di prenderci in castagna sul Senato federale, dicendo che bocciammo quella riforma del centrodestra che lo prevedeva. Non ci sono scorciatoie, però, presidente Gasparri: noi votammo contro quel modello di Senato federale, ma non illustro la storia precedente, il vostro voto in Bicamerale sul Senato federale e sulla riduzione del numero dei parlamentari, la fine ingloriosa della stessa

l'occasione per ringraziare ora - cosa che dimenticai di fare allora - il relatore Azzollini che ha condotto con grande scrupolo e grande intelligenza questa vicenda parlamentare. E io consento, naturalmente: il PdL voterà a favore; magari è contrario al Senato federale, però voterà a favore. Ma io vedo in questo un sintomo di quella indifferenza

come se il prezzo che oggi si paga con il federalismo fiscale assolvesse da qualunque altra condivisione di fondo. che non paghi perché, alla fine, questa indifferenza, attenta solo a ciò che onestamente si dichiara convenire, essere propria convenienza, rivela un'altra cosa: questa fortissima tentazione (più che una tentazione, direi) verso un modello autocratico, autocratico, tutto orientato alla mera convenienza, tutto orientato al rafforzamento del potere di uno. Esattamente il contrario della filosofia del federalismo fiscale e di quell'idea di governo dell'Italia. Ci preoccupa questa indifferenza, ma ci preoccupa soprattutto perché crediamo che non convenga al Paese.

senatori, voglio partire anch'io, come altri colleghi, dal rivolgere il mio ringraziamento al relatore, ai presidenti di Commissione Baldassarri, Azzollini, Vizzini, che in questi mesi molto hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo, a tutti i colleghi delle Commissioni, ai rappresentanti del Governo, numerosi, e, tra i tanti, ai ministri Calderoli e Fitto che fin dall'inizio hanno dato un contributo di passione e di competenza.

dello Stato unitario. Non ci sono parti del territorio che resteranno abbandonate. Non avremo però più amministrazioni in cui si spende a piè di lista, ma avremo amministratori che dovranno procurarsi le entrate e valutare con maggiore attenzione il livello delle spese. Vogliamo uno Stato più moderno e questa legge è il primo grande banco di prova di questa legislatura, approvata - come è stato ricordato - dopo un anno dall'insediamento del presidente Schifani e dall'avvio del nostro impegno di legislatori. Questa legge ci consentirà di razionalizzare la spesa, di combattere gli sprechi, di garantire meccanismi di solidarietà all'interno dello Stato. È una sfida che anche il Sud accetta ed affronta con determinazione. contiene norme che riguardano il Sud, dalla città di Reggio Calabria alle Regioni a statuto speciale, a tanti territori del Mezzogiorno che trovano risposte importanti. Vogliamo più velocità nelle istituzioni. il Popolo della Libertà, con la Lega, ha sottoscritto un patto politico che oggi raccoglie ancora più di ieri il consenso della maggioranza degli italiani. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Ed è in ragione di tale patto che oggi giungiamo a questo traguardo. Con la maggioranza degli italiani andremo avanti in queste scelte fondamentali. Voglio ricordare che questa non è una legge di alcuni contro altri, non è il federalismo del Nord contro il Sud.

Prendiamo atto però, nel contempo, del ruolo propositivo dell'opposizione, che anche oggi è emerso in tanti aspetti e in tanti interventi, e non lo sottovalutiamo. Ci auguriamo di poter lavorare insieme con lo stesso spirito nella Commissione bicamerale che sarà chiamata ad approvare i decreti di attuazione. Abbiamo voluto insieme una Commissione bicamerale proprio perché questa legge nasce in Parlamento, appartiene al Parlamento e il Parlamento dovrà attuarla, farla vivere e renderla una grande risorsa per tutta la Nazione. Dovremo andare avanti per valorizzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali, lo sviluppo delle aree a minore crescita e semplificare il sistema tributario; meglio sarebbe stato, colleghi se oggi aveste approvato quell'ordine del giorno del presidente Baldassarri che impegna ad affrontare con maggior vigore, fin dal prossimo DPEF, i temi della riforma fiscale. Completeremo questo lavoro con il codice delle autonomie locali, che sarà una tappa importante che affronteremo già dalle prossime settimane. Vogliamo ricordare in questa legge il fondo perequativo per le Regioni con maggiore capacità fiscale; perché questo è un federalismo che si collega ad un principio di sussidiarietà, al riconoscimento dei corpi intermedi e al rispetto delle comunità locali. Vogliamo insomma mettere un po' di ordine in quella riforma disordinata del Titolo V della Costituzione che la sinistra fece in fretta e con maggioranze risicate. Cominciamo a fare una riforma vera dello Stato, non le riforme con tre voti di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Anche l'esito della votazione di oggi dimostrerà la nostra maggiore saggezza. È giusto fare riforme insieme, ma deve essere un atto di volontà politica. La ricerca di convergenze non può nascere da ostruzionismi o da impedimenti ad un processo riformatore che il Paese da troppo tempo attende e del quale ha bisogno.

Non ci si faccia ingannare» - prosegue Panebianco - «dalla forza che concentra in sé oggi il *premier* Berlusconi: si tratta di una forza che ha ragioni politiche, non istituzionali». La Costituzione è quella dei governicchi, era quella delle crisi ogni sei mesi: è la forza del Governo e della maggioranza che dà stabilità al Paese, ma servono riforme per rendere permanente tutto ciò. Vogliamo quindi dire di sì al concorso delle volontà, ma diremo di no a un diritto di veto che condannerebbe all'immobilismo. La Costituzione si può cambiare: non è un totem ed è il capitolo ulteriore dopo questa sfida importante sul federalismo fiscale. Fermi i princìpi fondamentali, si possono introdurre innovazioni. Pietro Calamandrei disse: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé.

Noi vogliamo mettere, quindi, il combustibile del federalismo, il combustibile del presidenzialismo, il combustibile di una nuova Costituzione per la Repubblica italiana. Quando arrivarono al termine i lavori dell'Assemblea costituente, Meuccio Ruini, Benedetto Croce e lo stesso Calamandrei dissero che si sarebbe presto giunti ad un tempo in cui la Carta Costituzionale sarebbe stata necessariamente riformata. Ecco perché, approvando questa legge ordinaria, guardiamo già al traguardo di una riforma costituzionale che è anticipata, appunto, da questa legge. Il 7 gennaio 1981, intervenendo al comitato centrale del Partito comunista italiano, di cui era allora uno degli esponenti più autorevoli, Giorgio Napolitano affermava: si deve giungere ad una svolta effettiva nei metodi di governo, nel modo di concepire ed esercitare il potere, nei rapporti tra partiti, Stato e società, riaffermando pienamente i princìpi e le linee della Costituzione e ponendo mano a riforme e misure capaci di garantire il corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni. Ventotto anni fa, l'attuale Presidente della Repubblica, che nel Partito comunista italiano era una delle menti più aperte alle riforme, riconosceva inequivocabilmente la necessità di adeguamenti e ammodernamenti della nostra Costituzione. Gli storici discorsi di Croce e Calamandrei, che prima ricordavo, andrebbero riletti oggi con attenzione, di fronte al tentativo di affermare il principio antistorico e antigiuridico del dogma della immutabilità della Costituzione, secondo il quale chi vuole aggiornare alcune parti del nostro testo fondamentale sarebbe una sorta di sovvertitore della democrazia. Cari colleghi (e rispondo anche alla presidente Finocchiaro, al di là delle schermaglie su Senati federali o meno), la difesa e il rispetto dei princìpi fondamentali della Costituzione non implica l'immobilismo per quanto riguarda la seconda parte della Carta. I nemici della democrazia sono coloro che negano le riforme, perché uno Stato obsoleto, non in sintonia con le esigenze dei cittadini, finisce per delegittimarsi. Una democrazia, se opportunamente riformata, invece si rafforza. Il rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo ed altri capitoli andranno affrontati con coraggio e con spirito innovativo: ed è quanto vogliamo fare. Noi siamo lieti che su questo testo si sia realizzata una convergenza più ampia e siamo pronti ad accettare, sul terreno delle ulteriori e più importanti riforme, l'esigenza del confronto. Ribadisco, siamo disposti a subire i veti dell'immobilismo. Noi faremo le riforme in questa legislatura non lo hanno detto solo i Padri costituenti che mi sono permesso di ricordare né lo diceva, circa trent'anni fa, solo Giorgio Napolitano, ma lo dice la realtà della Costituzione materiale, quella che gli italiani vivono ogni giorno con una democrazia diretta che si è affermata fortemente, con una democrazia dei territori che è cresciuta con l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti delle Regioni. Quindi, con questa legge sul federalismo fiscale, noi facciamo partire la stagione delle riforme e speriamo, cari colleghi, di essere in tanti al traguardo. Il Popolo della Libertà ci sarà con la maggioranza degli italiani.

Signor Presidente, signori Ministri, responsabili del Governo, egregi senatori, voglio esprimere con questo intervento un voto di dissenso dal mio Gruppo e a nome **dell**'**Union** **Valdôtaine** e della maggioranza regionalista valdostana dichiarare un voto favorevole al disegno di legge. Prima di tutto per un giudizio positivo verso un percorso federalista, che oggi inizia anche per lo Stato italiano e che noi abbiamo già sperimentato, come utile e fondamentale per lo sviluppo, in più di 60 anni di esperienza autonomista. Votiamo nuovamente sì, come nel precedente passaggio al Senato, ma confermati in questo giudizio dalle modifiche apportate al testo nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati e che tengono conto delle osservazioni fatte dalle autonomie speciali (e di questo ringraziamo il ministro Calderoli). L'articolo 27, infatti, non prevede più, nella nuova formulazione, il patto di convergenza per le Regioni autonome, norma che avrebbe comportato contrasti con quanto prevede il nostro Statuto. positivamente che in quattro articoli del testo siano richiamati i territori montani come sede di attenzione specifica. Questo passaggio sarà fondamentale per determinare i nostri costi standard; anche se, signor Ministro, bisognerà definire cosa si intende per montagna. Con il voto positivo esprimo, comunque, il disappunto per la recente dichiarazione di un Ministro di questo Governo contro le autonomie speciali, ritenendo oggi che queste dichiarazioni siano state espresse solo a titolo personale. Anche per questo vigileremo sulla realizzazione della riforma che oggi verrà approvata, chiedendo al Governo nei passaggi successivi rapporti chiari e precisi. Signor Presidente, da qualche tempo la religione politica in auge nel nostro Paese ha sancito una sorta di undicesimo comandamento, quello che prescrive all'Italia di diventare tutto ad un tratto un Paese federale. Vorrei sommessamente segnalare ai cultori di questo credo, di cui non faccio parte, che la rigorosa osservanza di questo comandamento richiederebbe semmai di partire dalle regole e non dalle risorse, dal federalismo istituzionale e non da quello fiscale e soprattutto richiederebbe, almeno di questi tempi, di non moltiplicare i centri di spesa. Con il voto di oggi si vorrebbe inoltre aggiungere un dodicesimo comandamento, quello che impone all'opposizione di partecipare gioiosamente a questo voto, senza conoscere né il costo economico, né le conseguenze istituzionali del consenso che con la nostra astensione siamo chiamati ad esprimere. Non voglio turbare il clima di dialogo che da qualche giorno spira nella politica italiana, temo però che questo dialogo nasconda un equivoco: infatti, se questa legge verrà attuata, salterà la spesa; se questa legge non verrà attuata, salterà l'alleanza di governo. Per superare questa contraddizione temo che si stia facendo saltare il senso comune. Per queste ragioni il mio voto sarà contrario.